L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun Gruppo ha a disposizione 20 minuti, comprensivi degli interventi in discussione generale ed in dichiarazione di voto.

per responsabilità e nella consapevolezza della situazione di emergenza in cui ci troviamo, che è sotto gli occhi di tutti, non per propaganda o tanto meno

di carattere più generale ed organico, vedi la riforma degli ammortizzatori sociali, di cui da tanto tempo, troppo, si parla e che tutti abbiamo trascurato. Tra l'altro, le avanziamo con urgenza perché nella situazione italiana, che risente della gravità mondiale, vi è in più una carenza, una grave difficoltà. L'Italia è l'unico dei grandi Paesi europei che non ha una rete di sicurezza, quale un sistema universale di sostegno a chi sta per perdere il posto di lavoro e a chi lo ha già perso. Questo ci mette tutti in difficoltà, il Paese ed i singoli, perché avere una simile rete di protezione non è solo un atto di giustizia e di sostegno alle persone, ma anche un grande stabilizzatore economico e sociale, come tutti sanno e richiedono. avere questa consapevolezza è fondamentale e ci sorprende che la nostra proposta sia stata accolta come una improvvisata voglia di pubblicità. Le proposte sono due: la prima, di cui si è parlato di più, è quella dell'introduzione, in via eccezionale per quest'anno ma nella prospettiva di una riforma generale, di un assegno mensile per i disoccupati, per tutti quelli cioè che perdono il posto di lavoro. Questa richiesta si spiega proprio per quanto detto prima. Attualmente solo una parte dei lavoratori che perde il posto di lavoro gode di una tutela del reddito. Questo è inaccettabile.

purtroppo, hanno perso o stanno per perdere il posto di lavoro è urgente che tutti abbiano un sostegno, che noi indichiamo nella misura comune per i disoccupati già tutelati. I dati sono chiari. Facciamo un atto di giustizia ed estendiamo a tutti quello che solo alcuni hanno.

in passato. In quelle situazioni in cui una crisi temporanea mette a rischio la tenuta delle imprese, la cassa integrazione temporanea permette di sostenere i lavoratori senza gravare sui bilanci delle imprese, soprattutto le piccole, che sono prive di questo sistema e che, se non glielo riconosciamo, rischiano di chiudere anche quando sono sane e rischiano di fare

licenziare. Questa è veramente un'inaccettabile falsità, perché il sistema di prevenzione va rafforzato e generalizzato in quanto anche la cassa integrazione non è prevista per gran parte delle piccole imprese; è chiaro che se poi la crisi

Signora Presidente, come Italia dei Valori abbiamo deciso di presentare questa mozione e quindi di chiedere alcuni impegni al Governo, preso atto oggettivamente di come la crisi finanziaria internazionale si sia ormai trasformata in una crisi economica pesante anche nel nostro Paese. Peraltro, diversi istituti di previsione, la Banca d'Italia e la Confindustria, ci dicono che per il 2009 le previsioni non sono rosee: è prevista infatti una caduta del PIL superiore al 2,5 per cento e un aumento della disoccupazione sopra l'8

nostra economia, a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e parasubordinati occupati in quelle aziende che rinuncino alla cassa integrazione ma che riducano gli orari di lavoro, a fronte della riduzione degli ordini. Quindi, una sorta di contratto di solidarietà. poi una riforma più complessiva della cassa integrazione e degli ammortizzatori sociali. In questa mozione, com'è compito di una forza politica seria, indichiamo ovviamente anche dove andare a prendere le risorse per poter sostenere finanziariamente

in una riduzione dei costi della politica e degli sprechi della pubblica amministrazione, andando, per esemplificare, ad una riduzione dei rimborsi elettorali e degli stipendi, altissimi talvolta, dei manager della pubblica amministrazione, e alla soppressione di enti inutili;

come si direbbe, a stretto giro di posta, misure che potessero concretamente portare avanti quei princìpi e quelle indicazioni che la

delle piccole e medie imprese, quali la semplificazione amministrativa, la capitalizzazione delle imprese, la facilità di accesso al credito e il sostegno alla crescita dimensionale delle imprese.

fortissima e improrogabile di ridurre i tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese. Nel 2008 siamo arrivati a 839 giorni di ritardo nei pagamenti. Questa è una situazione intollerabile che strangola le piccole e medie imprese e che le costringe spesso a

la mozione che presentiamo scandisce le linee d'intervento economico-sociale del Governo di fronte all'alluvionale irrompere della grande crisi. Credo vada doverosamente sottolineato come i presupposti stessi su cui si fonda la linea d'intervento del Governo siano radicalmente altri rispetto a quelli su cui si fonda la proposta di intervento nella medesima materia dei colleghi dell'opposizione. Sono due modi radicalmente diversi di intendere le origini della crisi e, dunque, i modi per affrontarla, per risolverla e per uscirne. È una crisi da domanda quella che sta gravando sul Paese, non una crisi da offerta. Ed ecco allora che le proposte, soprattutto dei colleghi del Partito Democratico, funzionali da un lato a rafforzare il *downsizing* (il ridimensionamento delle imprese per consentire loro il miglioramento della struttura dei costi affinché siano più agili nell'affrontare una sfida competitiva), sono sbagliate perché non c'è nessuna sfida competitiva in atto generata da una condizione di deficit sulla struttura dei costi, ma esiste invece una crisi da domanda.

In qualche modo sembra ricomparire - e mi dispiace dirlo - nell'opposizione una cultura attardata su modelli novecenteschi. È in qualche modo novecentesca questa ossessione demiurgicamente pianificatoria, questa vocazione allo sdrucciolamento nell'antagonismo così giacobino, così savoiardo, così conflittuale. *(Brusìo).* PRESIDENTE Colleghi, scusate, già

un'idea ancora antagonista della società, ancora pianificatoria dei mezzi per affrontare e sciogliere l'antagonismo. Lo ripeto, è una soluzione novecentesca. Nello stesso tempo, va accuratamente evitata ogni azione che generi e determini una condizione di insicurezza, anche psicologica, nel governo della crisi. Sotto questo profilo, ad esempio, appare particolarmente incauta la proposta di intervento di tassazione sui redditi più alti perché, proprio nel momento in cui si appalesa una crisi da domanda e quindi il consumo andrebbe agevolato, chi

Un altro tema va affrontato con molta limpidezza. Noi non possiamo immaginare in questa fase riforme strutturali degli ammortizzatori sociali, perché questa crisi è completamente nuova.

di salvataggio del mondo attraverso quelle riforme strutturali che, invece, corrono il rischio di essere ideologicamente raggrumate in se stesse o prigioniere di un'incapacità di lettura autentica, dinamica e propulsiva della realtà economica del Paese. Sotto questo profilo, ancora, il comportamento del Governo è funzionale ad intervenire su una crisi (che è crisi da domanda e non da offerta) e a mantenere vivace, vivace, continuativo e pronto alla ripartenza il collegamento tra la condizione professionale e la condizione d'impresa. È un comportamento pragmaticamente attento al delinearsi di una crisi i cui contenuti non si sono ancora tutti appalesati e dispiegati e rispetto ai quali bisogna tenere forze tenere forze fresche di riserva, pronte ad essere collocate in una battaglia che oggi non è ancora quella decisiva. I 100 trilioni di dollari che hanno generato l'asfissia del sistema economico mondiale potrebbero infatti conoscere altre varianti rispetto alle quali dobbiamo essere pronti ad intervenire. Questa mozione del Popolo della Libertà, che il Governo sostiene insieme agli alleati della Lega Nord, che danno un contributo collegato alla loro capacità dinamica di atteggiare risposte anche rispetto alle loro concrezioni territorialmente dispiegate, è a nostro avviso l'unica in grado di segnare un orizzonte positivo in questo momento così arduo per il Paese.

durissima dal punto di vista economico e sociale ma che ha delle specificità e delle peculiarità. lo sforzo complessivo del Governo, che ovviamente si sta ancora dispiegando, per trovare differenti strumenti di sostegno di sostegno rispetto alle diverse emergenze: da quelli che concernono strettamente il sistema degli ammortizzatori sociali, a quelli riguardanti il sostegno alle banche per non interrompere il credito alle imprese e alle famiglie, allo stimolo all'economia produttiva attraverso grandi investimenti nel settore infrastrutturale. Abbiamo apprezzato anche lo sforzo di raccordo e di concertazione con le parti sociali, sintetizzato nel protocollo di febbraio.

viene meno all'attenzione rispetto al territorio meridionale. Infatti, il complesso di queste manovre, che guardano al sistema economico complessivamente, manca, secondo noi, di un'attenzione e di una sensibilità particolare rispetto Il nostro - mi dispiace doverlo ribadire con questa sorta di cantilena che spero non annoi - è un Paese spaccato, un Paese duale, sia per quanto concerne la qualità dei servizi, sia per quanto concerne la consistenza della sua dotazione infrastrutturale, ma anche nella sua trama produttiva. Il sistema produttivo meridionale, caratterizzato da piccole e piccolissime imprese, da strutture artigianali, da dimensioni familiari, rimane estraneo al meccanismo tradizionale degli ammortizzatori sociali concepiti correttamente nella cultura dell'economia fordista per la grande industria privata nazionale. È un problema serio, che si pone in termini di giustizia e di equità, anche perché le Regioni meridionali hanno concorso a definire la consistenza economica delle risorse che che vengono utilizzate dal Governo per contrastare la crisi e vi è bisogno di misure mirate in termini di flessibilità perché si riesca a contrastare i meccanismi i meccanismi della inoccupazione e della disoccupazione che in questo momento stanno caratterizzando anche l'area del precariato, che nel Sud è particolarmente sviluppata, quindi con una politica di assoluta attenzione. con la nostra mozione, che il Governo calibri le riposte, che sappia concepire delle misure flessibili, che intervengano anche a tutelare queste aree di particolare debolezza, utilizzando anche la utilizzando anche la possibilità che la Cassa depositi e prestiti e le risorse disponibili vengano impegnate, attraverso accordi di programma quadro con le Regioni, per intervenire sulle emergenze imprenditoriali, oltre che con un meccanismo di

Ho sentito il Ministro dell'economia considerare le pensioni un ammortizzatore sociale, ma è necessario affrontare il tema di una profonda rimodulazione del sistema previdenziale italiano per trovare risorse nuove e più flessibili che riguardino aree diverse rispetto al tradizionale Il sistema previdenziale italiano è un sistema vecchio, che va rimodulato perché deve liberare risorse per una politica dello sviluppo seria e per una politica di sostegno sociale assolutamente più flessibile.

*(IdV)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, i dati che vengono resi noti ogni giorno riguardo gli effetti di questa crisi, soprattutto sull'occupazione, sono veramente preoccupanti e richiedono un intervento incisivo. Sono di alcuni giorni fa i dati dell'INPS secondo cui, nei soli primi due mesi del 2009, i disoccupati che hanno fatto domanda del sussidio di disoccupazione in Italia sono stati 370.561, con un incremento del 46,13 per cento rispetto allo scorso anno. Dati comunque parziali, in quanto non registrano il numero di tutti coloro che non hanno diritto all'indennità e che, purtroppo, sono destinati a crescere dato che a luglio scadranno quasi un milione di contratti a termine e nel secondo semestre del 2009 se ne aggiungeranno un altro milione e Per non parlare di quello che accadrà a breve a molti dei lavoratori precari della pubblica amministrazione che, se verrà approvato l'articolo 7 del collegato sul lavoro alla finanziaria, vedranno svanire, dopo anni di lavoro, ogni possibilità di stabilizzazione e, addirittura, di rinnovo del contratto. Non abbiamo ancora dati ufficiali aggiornati, ma il numero dei precari della pubblica amministrazione a fine 2007 era di circa 200.000 lavoratori, senza contare i 240.000 nominativi delle graduatorie ad esaurimento della scuola. I lavoratori precari in Italia rappresentano il 12 per cento dell'occupazione totale, milioni di lavoratori con un contratto tipico di quella che una volta si chiamava flessibilità. Noi dell'Italia dei Valori crediamo nella libera impresa e crediamo che l'impresa, in un'economia di mercato, si possa fare solo a condizione che vi sia anche flessibilità del lavoro, ma la realtà è che la flessibilità è stata sostituita oggi, purtroppo, dalla precarietà. È per questo che riteniamo fondamentale una riforma profonda degli ammortizzatori sociali, da concordare con tutte le parti in causa, che preveda, soprattutto a fronte di questa crisi, un'indennità di disoccupazione tale per cui venga garantito a tutti i lavoratori, con qualsiasi tipologia di contratto, il mantenimento del reddito in caso di perdita o assenza del lavoro. Inoltre, per fare in modo che, nonostante la crisi delle imprese, quanti più dipendenti conservino il posto di lavoro, riteniamo necessario che si facciano degli interventi affinché le aziende, modulando gli orari di lavoro in base al nuovo ridotto livello produttivo, stabiliscano un monte delle retribuzioni con una riduzione dei compensi erogati dal datore di lavoro per la diminuita attività lavorativa da compensare attraverso gli ammortizzatori sociali. Questo è il senso della nostra mozione. Si tratta di un intervento simile a quello proposto in Germania dalla cancelliera Merkel, che mira a permettere alle imprese di poter continuare la propria attività (sia pure ad orario ridotto) senza far perdere ai lavoratori i redditi percepiti prima dell'inizio della crisi e che, quindi, sostiene i redditi delle famiglie. Ovviamente questo dovrà essere un intervento temporaneo, riservato a quelle imprese che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione e che sottoscrivano un impegno a non diminuire i dipendenti per 24 mesi, a ridurre al minimo l'eventuale esternalizzazione all'estero della produzione, e che siano, ovviamente, in regola con gli obblighi fiscali. Se non si sostengono i redditi dei lavoratori sarà difficile riprendersi da questa crisi, in quanto le mancate entrate hanno già e avranno conseguenze sui consumi, che calano e caleranno ulteriormente, e questi sulla produzione delle aziende, in un corto circuito dell'economia da cui sarà difficile uscire. Se si vuole davvero affrontare questa crisi, e trovare soluzioni, è necessario, come sta accadendo negli Stati Uniti, voltare pagina. Prendiamo esempio dal presidente Obama, che nei prossimi tre anni raddoppierà la quota di energie rinnovabili, creando così nuovi posti di lavoro e rimettendo in moto l'economia, nel rispetto dell'obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra. In Italia, come già sta accadendo negli Stati Uniti, è necessario coniugare sviluppo e ambiente, puntando su nuove tecnologie che ci permettano di competere con le sfide del mercato globale di assolvere ai doveri di efficienza energetica, imposti anche dall'Unione europea, prevedendo investimenti nelle energie rinnovabili per creare occupazione e risparmiare energia, investimenti nelle tecnologie pulite per rilanciare i settori dell'edilizia e dell'industria automobilistica, investimenti nelle infrastrutture e nell'interconnessione per promuovere l'efficienza e l'innovazione. Le misure previste fino ad oggi dal Governo si sono rivelate inefficaci, delle elemosine: basti vedere la vicenda della *social* *card*, a cui, peraltro, neanche tutti gli aventi diritto sono riusciti ad accedere. È ormai evidente che questo Governo ad oggi non ha risposto efficacemente a questa crisi che sta mettendo a dura prova i lavoratori e le loro famiglie. Invito, pertanto, tutti i colleghi a votare per la nostra mozione perché i dati parlano chiaro. Abbiamo il dovere di rispondere subito a 11.500 interinali, 25.213 lavoratori socialmente utili, 112.489 lavoratori con contratto a tempo determinato, 4.315 giovani entrati nella pubblica amministrazione con contratto di formazione lavoro e, per finire, 58.536 con contratto

Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Paese sta indubbiamente attraversando una delle crisi peggiori degli ultimi 80 anni. La gravità della situazione ci impone l'adozione di interventi strategici

che ci impone di avviare una nuova politica economica che sia al fianco delle famiglie e delle imprese, per metterle al riparo anche dai rischi della finanza virtuale e da quella speculativa, che tanti danni hanno arrecato. A questo punto è necessario, se non strategico, tornare ai valori tradizionali dell'economia, basata sui beni e sui servizi che vengono prima del denaro. Centrale in questa prospettiva è il ruolo delle imprese, in particolare delle piccole e medie realtà produttive, che costituiscono la vera ricchezza del nostro Paese. Senza la fatica di tante imprese artigiane o piccoli industriali, che hanno reso grandi i nostri marchi anche all'estero, non avremmo infatti potuto raggiungere quell'eccellenza che ci contraddistingue in molti ambiti produttivi. L'incontro di ieri sera tra il presidente Berlusconi e i banchieri e l'iniziativa del ministro Maroni per l'accesso al credito di imprese e famiglie sono un buon inizio per poter ridare la fiducia necessaria al rilancio della nostra economia. Le banche, infatti, devono essere responsabilizzate nella costruzione di un nuovo ruolo di effettivo all'economia, evitando il taglio generalizzato delle linee di credito, che produrrebbe la morte delle piccole e medie imprese. In questa delicata situazione, il primo problema che da affrontare è l'occupazione, dove al Nord, in Padania, sta registrando una fase negativa e una contrazione, per cui è necessario assolutamente intervenire. I nostri lavoratori non devono essere lasciati soli. Vi abbiamo già in larga misura provveduto in larga misura provveduto grazie a interventi varati o programmati dal Governo a sostegno degli ammortizzatori sociali. Sono misure che riguarderanno tutti i lavoratori, anche quelle atipici. Solo con questa strategia di intervento possiamo effettivamente rilanciare l'economia del Paese. Non condividiamo le misure proposte dall'opposizione, incentrate su una politica prettamente assistenzialistica. Tali interventi infatti rischiano di rappresentare un costo per lo Stato, senza risorse per il sistema produttivo. La vera risorsa sono i lavoratori che, insieme agli imprenditori e agli artigiani, stanno faticando non poco a tenere dritta la schiena per non far crollare il sistema produttivo e a questo la Lega Nord tiene molto: difenderemo con i denti il lavoro inteso come vero rilancio per superare questa crisi. Oltre a responsabilizzare le imprese attraverso incentivi e aiuti economici, anche rivolti ai lavoratori, è indispensabile stare al fianco delle famiglie per aiutarle a sostenere i consumi, a poter spendere in modo che il volano economico ricominci a girare. Le famiglie sono ancora i primi, autentici ammortizzatori sociali del nostro sistema produttivo. Sconfiggere la disoccupazione che produce contrazione nei consumi, rilanciare le imprese e l'artigianato con adeguate misure cui devono essere partecipi sia il mondo bancario sia quello politico e istituzionale: tutto questo impone un grande lavoro cui dobbiamo dedicarci con passione e con amore; amore per il bene delle nostre famiglie, dei nostri lavoratori e della nostra economia. Solo così possiamo offrire risposte effettive a questa crisi generalizzata.

e dell'irresolutezza e dell'incapacità dell'azione del Governo e del Parlamento a produrre risposte adeguate ed organiche per affrontare una crisi, il cui carattere emergenziale ha ormai sempre più a che fare con le sue proporzioni,

si snoda intorno a due temi cruciali: tutelare e cambiare. La tutela riguarda innanzitutto il patrimonio produttivo del Paese, fatto di grandi imprese industriali, ma soprattutto di piccole e medie imprese, di imprese artigiane e commerciali, di cooperazione, di attività produttive anche individuali. Molte di queste realtà rischiano la chiusura, o quantomeno la perdita del loro principale strumento produttivo - il capitale umano - se non saranno accompagnate nella fase, che speriamo temporanea, ma sappiamo essere lunga, di contrazione dell'attività, da ammortizzatori sociali efficienti e efficaci che consentano loro di rimodulare l'attività, di sospenderla temporaneamente, senza perdere il legame organizzativo con le proprie risorse professionali. Molte di queste realtà, per dimensione o per settore produttivo, ma anche per le tipologie contrattuali a cui hanno fatto ricorso negli ultimi anni (si veda, ad esempio, il dato delle imprese del Nord-Est, che hanno incrementato l'occupazione dei cosiddetti contratti precari di oltre il 25 per cento negli ultimi cinque anni) sono escluse dall'accesso agli ammortizzatori sociali, anche da quelli in deroga. C'è la necessità di prevedere, quindi, nuove e più adeguate tutele in presenza di riduzione dell'occupabilità innanzitutto per le imprese che hanno più ampiamente ampiamente contribuito allo sviluppo del Paese. Di questa necessità ci hanno dato conto le rappresentanze imprenditoriali che abbiamo ascoltato in questi mesi in Commissione lavoro nel corso delle audizioni sul collegato alla finanziaria. Ci hanno detto che c'è bisogno di nuovi ammortizzatori sociali per non chiudere, per andare avanti. L'altro tema della tutela riguarda i redditi da lavoro delle persone, delle famiglie, delle donne e dei giovani e con esso la tutela del tessuto sociale, la tenuta della convivenza civile nel nostro Paese. Abbiamo lungamente discusso in Aula dei dualismi che lo caratterizzano, che caratterizzano, in sostanza, il nostro *welfare*. Quello tra lavori tutelati e non tutelati rappresenta senz'altro la divaricazione principale in quest'ambito; al suo interno, però, ce ne sono altre: quella tra donne e uomini, di cui abbiamo lungamente discusso ieri, purtroppo (lo dico

e i 600.000) lo perderanno per analoghe ragioni, in quanto titolari dei contratti a termine nel corso del 2009. Tutti costoro non hanno accesso ad alcun sostegno economico; non mi sento infatti di qualificare come sostegno economico effettivo la provvidenza prevista dal decreto-legge

La proposta contenuta nella nostra mozione intercetta questi bisogni (e altri di profilo analogo) e fornisce una risposta immediata, da rendere operativa entro il 31 marzo, a migliaia di piccole e medie imprese e a centinaia di migliaia di persone e di famiglie.

In questo momento occorre spendere meno, spendere meglio e pagare tutti. E l'attuale sistema degli ammortizzatori è squilibrato, perché gli ammortizzatori in deroga sono per larga parte, anzi per la totalità, in carico alla fiscalità generale. l'ultimo punto della nostra proposta - procedere ad una riforma complessiva degli ammortizzatori, che è tanto più necessaria in questo momento proprio

ma, al contrario, significa pianificare, verificare, e rimodulare sulla base dei risultati della verifica. Una riforma strutturale, in senso universalistico può consentire di superare, per il futuro, ogni profilo assistenzialistico, garantendo universalità all'interno di un sistema integrato e proattivo in direzione di un obiettivo comune, quello del miglioramento delle condizioni di sviluppo dei singoli e del sistema economico e sociale del nostro Paese.

non pretendendo certo di avere l'unica soluzione, né tantomeno una soluzione che possa essere accettata unanimemente. Vogliamo riportare il tema della crisi economica e sociale dal livello del dibattito economico, o ancora peggio mediatico, perché il Parlamento, in queste circostanze, deve assumere il ruolo che gli compete, sapendo che, alla fine, il Governo dovrà assumersi ogni responsabilità politica e morale su questo grande tema. Noi vogliamo essere realisti: la crisi finanziaria globale, a detta di molti, appare ancora lontana dalla soluzione, mentre i suoi effetti sull'economia reale cominciano, con scenari che cambiano e si aggravano di giorno in giorno, a dispiegarsi in tutta la loro virulenza e drammaticità. Il mondo del lavoro, con il fronte delle tutele sociali, sta rischiando sempre di più di sprofondare in questa crisi. Negli ultimi due mesi, più di 372.000 lavoratori hanno perso il posto e chiesto l'indennità di disoccupazione. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, abbiamo avuto un aumento del 46 ma sono dati purtroppo solo parziali, che riguardano solo coloro che possiedono i requisiti per ricevere l'indennità. Sappiamo, infatti, che i due anni di iscrizione all'INPS le 52 settimane di contributi sono criteri che tagliano fuori un pezzo consistente del nostro Paese, un pezzo consistente di nuovi disoccupati, quelli con i contratti atipici, dal tempo determinato ai contratti a progetto. Per essere più chiari e comprendere sino in fondo l'entità della piaga del lavoro che non c'è, poco più di una settimana fa (parliamo di 7-10 giorni fa) il commissario José Barroso

Noi vogliamo essere responsabili. Sappiamo benissimo che la recessione europea e mondiale non può essere certo fermata per il momento:

Agli italiani interessa poco il dibattito su quante e quali *bad bank* siano da costituire, su come i titoli tossici saranno tolti dai bilanci delle banche; banche; interessa molto di più mettere al centro delle risposte alla crisi la difesa dei redditi più bassi, la garanzia al sostegno delle piccolo e medie imprese, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali. Ci sono almeno due questioni che potrebbero e dovrebbero essere sciolte: la prima che cosa dire agli italiani, la seconda che cosa fare al più presto. Sulla prima dobbiamo prendere atto che il Governo continua in una sua personale strategia comunicativa finalizzata a ridimensionare gli effetti della recessione e a rassicurare sulla idoneità degli strumenti messi in campo, sui quali abbiamo avuto più volte occasione di esprimere le nostre perplessità. prima il Capo del Governo dichiara che la crisi c'è, ma non è grave; poi aggiusta il tiro e dice che la crisi è grave, ma senza miseria. il profilo strategico delle politiche economiche e sociali sta assumendo i connotati, per usare un rispettoso eufemismo, del paradosso politico: inizialmente, la proposta di detassazione degli straordinari, poi abbandonata; la proposta della settimana corta, anch'essa abbandonata. Si tratta di atteggiamenti schizofrenici che promettono l'estensione delle tutele e, di fatto, smantellano e smontano quelle esistenti. Il piano anticrisi in due tempi, che risale solo ad alcuni mesi fa, con i 500 milioni di euro per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga e con la proroga di sei mesi per l'attuazione delle deleghe, ereditata dal precedente Governo per riformare gli ammortizzatori sociali, riordinare le normative sui servizi all'impiego, sull'apprendistato e sull'occupazione femminile, si è dimostrato del tutto inadeguato. È vero che la crisi è la più complessa dell'ultimo mezzo secolo; è vero che essa cambia forma e sostanza di giorno in giorno, al punto che la tanto decantata *Robin tax*, che risale soltanto al mese di luglio, acquista un valore di ridicola preistoria; è vero che costringe i Governi a ripetuti aggiornamenti statistici e a continui interventi normativi, come dimostra la Nota informativa 2009-2010 sugli andamenti di finanza pubblica,

a conferma di un lassismo fiscale cui sembra ispirarsi l'azione del Governo e che abbiamo già avuto modo di discutere più volte, in quest'Aula. È certo, dalla crisi sta emergendo l'urgenza di un nuovo tipo di economia e di impresa. C'è una riforma, quella degli ammortizzatori sociali, che in Italia deve servire sia a ridurre i costi sociali della crisi che a permettere la conservazione del lavoro in settori in cui possiamo meglio reggere la concorrenza internazionale. Sappiamo che in Italia chi è disoccupato è dodici volte più a rischio di essere povero rispetto al resto della popolazione.

per cento del totale dei dipendenti italiani, escluso il pubblico impiego, non hanno alcuna misura di sostegno al reddito e, nel caso in cui la propria azienda, per le difficoltà economiche in atto, li allontanasse, si troverebbero senza garanzie e senza copertura salariale. un vero e proprio esercito di lavoratori invisibili perché, quando stanno a casa, non se ne accorge nessuno. Al vertice di questa classifica, vi sono i due milioni di lavoratori del settore dei servizi, gli occupati del commercio alle dipendenze di aziende con meno di 200 addetti, quelli dell'artigianato, quelli del settore delle Gli strumenti in deroga sin qui adottati stanno dimostrando tutti i propri limiti: innanzi tutto, si rivolgono alle imprese e non ai disoccupati; secondo luogo, sono uno strumento di politica industriale ed è quindi la politica a decidere discrezionalmente a quali imprese dare gli ammortizzatori; in terzo luogo, e non da ultimo, non istituiscono alcun diritto soggettivo ad essere aiutati quando si perde il lavoro. Questo significa, ed è il senso della nostra proposta contenuta nella mozione, che occorre soprattutto disporre di buoni ammortizzatori sociali, che devono integrare il reddito a fronte di una riduzione dell'orario di lavoro, senza che vi sia l'allontanamento del lavoratore, e devono consentire alle imprese di ridurre i costi del personale durante le fasi di contrazione della domanda, al fine di potersi ristrutturare in un periodo di tempo adeguato. Proponiamo la stipula di un contratto di solidarietà: non proponiamo l'acqua calda né nulla di nuovo, ma la stipula di un contratto di solidarietà, che comporta per i lavoratori la concessione del trattamento d'integrazione salariale, per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, evitando il licenziamento, l'allontanamento e l'estraneità dei lavoratori ritenuti in esubero. comporta, per i datori di lavoro, una riduzione dei contributi previdenziali assistenziali, conservando però le competenze, le professionalità ed il *know how* dell'azienda.

Salvare il Paese dalla crisi, ma soprattutto contrastare le nuove disuguaglianze sociali è un obiettivo ambizioso, tale da giustificare ogni sforzo: trincerarsi - come sta facendo il Governo - dietro alla scarsità di risorse economiche indica soltanto che non vi è alcuna volontà politica. Non è questione di tesoretti o di gruzzoletti come ha sottolineato il ministro Tremonti - né di avanzare proposte da apprendisti stregoni - come ha dichiarato il ministro Brunetta - ma solo di prendere piena consapevolezza, insieme alla crisi sociale, di due elementi. tutto, per favorire insieme il mercato e la giustizia distributiva è indispensabile, soprattutto in Italia, arricchire e migliorare gli ammortizzatori sociali; in una fase di profonde ristrutturazioni produttive gli aiuti per chi perde il posto di lavoro vanno messi a disposizione senza guerre tra poveri. In secondo luogo, la spesa pubblica in ammortizzatori sociali non contrasterà la recessione attuale, ma frenerà semmai la seconda fase recessiva e favorirà così la ripresa, appena sarà possibile.

Una modifica degli ammortizzatori sociali per ampliare il perimetro di riferimento a tutti i lavoratori porterebbe ad un aumento del disavanzo pubblico, che tuttavia sarebbe solo temporaneo, dato che andrebbe a riassorbirsi nella fase di congiuntura positiva. I tempi stringono: non basta aver fatto l'accordo da 8 miliardi tra Regioni e Governo, se non si fa in fretta e se non si dice come distribuire le risorse.

coperture debbono necessariamente esserci. Per questo chiediamo all'Aula di valutare e approvare questa nostra proposta: non è l'unica che può essere messa in campo, tant'è vero che voteremo con convinzione la mozione presentata dai colleghi del Partito Democratico, ma oggi si chiede al Parlamento una prova di responsabilità, di sensibilità e di compattezza, e di compattezza, non solo per dare una risposta concreta ai problemi degli italiani, ma soprattutto per riavvicinare le istituzioni al Paese. *(Applausi

il dibattito di oggi ha affrontato sicuramente l'aspetto più grave della crisi economico-finanziaria di questo Paese: la perdita di posti di lavoro. Ho sentito ipotesi di soluzioni diverse a questo problema, alcune molto interessanti e condivisibili, ma come donna del Sud, consapevole della particolare situazione di gravità in cui versa l'economia meridionale, devo condannare quello che ritengo il principale cancro della nostra economia: l'assistenzialismo. È da troppi anni che se ne fa uso e abuso. Dobbiamo trovare il coraggio di fermare una pratica che crea un circolo vizioso. Se si continua ad offrire solo assistenza, se ne chiederà sempre di più, anche perché al Sud, grazie al minor costo della vita, di assistenzialismo si può vivere, ma purtroppo, come è facile verificare, si può anche morire.

Infatti, fino ad oggi, il sistema assistenzialista ha provocato solo buchi neri, come ad esempio le folli spese sanitarie a fronte di servizi scadenti. Dobbiamo, invece, cercare di creare le condizioni affinché i giovani possano pensare al proprio futuro, rimboccandosi le maniche per lavorare,

Il nuovo modo di fare politica al Sud deve puntare allo sviluppo, a creare ricchezza da ridistribuire e non a ridistribuire solo quella che c'è, che non è tanta. Il Sud deve cominciare a portare avanti un progetto che permetta di avere una politica del territorio e un uso appropriato delle proprie risorse, con particolare Valorizzando e utilizzando adeguatamente le proprie bellezze naturali, paesaggistiche e culturali, il Sud potrebbe trovare la chiave del proprio riscatto. bisogna creare le condizioni per far emergere il lavoro nero, non creare altri posti di lavoro fittizi o socialmente utili, come invece una certa sinistra ha fatto negli ultimi anni.

in Robin Hood che tolgono ai ricchi per dare ai poveri. Certamente ci sono gli estremi, come i super ricchi e le fasce veramente bisognose, ma le politiche devono essere sensate. L'obiettivo primario deve essere lo sviluppo.

che bene o male ci mantiene, deve finire, altrimenti il Sud non crescerà mai. Ciò che salverà il Sud - non solo secondo me, che rappresento la Lega Nord,

Signora Presidente, abbiamo presentato una mozione che, a differenza di quella presentata dai colleghi del Partito Democratico, che rispettiamo, ha lo scopo di affrontare in termini più ampi il tema della crisi occupazionale ed economica del nostro Paese.

non è neanche dignitoso continuare in queste condizioni. Ci sono molti luoghi dove avviare colloqui, di cui certamente avete bisogno, ma non in Aula.

In realtà, il quadro di riferimento con cui dobbiamo fare i conti è obiettivamente preoccupante sia a livello mondiale, visto che si stima un calo drammatico della produzione industriale del 15 per cento, calo che non si avvertiva dai tempi della Seconda guerra mondiale nel sistema cosiddetto globale, sia con riferimento al contesto nazionale nel quale ci muoviamo, ove si consideri che la stima del PIL nel nostro Paese per cento per l'anno 2009 sui dati Bankitalia aggiornati rispetto alle stesse previsioni di gennaio, che davano una flessione del PIL per 2009 pari al 2 per cento ed una ripresa della crescita dello 0,5 nel 2010. In questo contesto, anche i dati che provengono da Confindustria, che certamente non ha interesse ad essere disfattista nel nostro Paese, né a non concorrere con tutti noi a produrre iniezioni di ottimismo e di fiducia

previsto, come noto, nella perdita di circa 600.000 posti di lavoro, con un livello della disoccupazione all'8,4 Questi dati sono confermati dal rapporto sulla protezione e l'inclusione sociale della Commissione dell'Unione europea ed evidenziano che in Italia probabilmente salirà ulteriormente il tasso totale delle persone a rischio povertà, un tema del quale dobbiamo occuparci. sostenuto la proposta, venuta dal segretario del Partito Democratico, sul contributo di solidarietà. Non lo riteniamo esaustivo di tutti i problemi, ma certamente è uno strumento che può dare un segnale forte di inversione di tendenza.

sottolineato anche dall'incremento pesante del ricorso alla cassa integrazione, con l'inevitabile crescita dei conti pubblici.

prima parte del 2009, nonostante si sia in presenza di sistemi economici, il nostro e quello americano, totalmente diversi e nonostante, obiettivamente, la nostra economia abbia manifestato segnali di reazione positiva rispetto agli Stati Uniti nei confronti della crisi. In questo contesto è evidente che le caratteristiche positive del nostro Paese vanno guardate con riferimento alla capacità crescente di risparmio delle nostre famiglie e delle imprese nostro sistema di piccole e medie imprese flessibile, capace di adattarsi alla più difficile situazione competitività determinata dalla crisi. È giusto e corretto ciò che in questo senso il Governo sostiene e cioè che una delle spirali negative è data dalla mancanza di fiducia e che, quindi, è necessario intervenire per infondere fiducia nel sistema. per alimentare la fiducia e per immettere iniezioni di speranza nel sistema economico del nostro Paese, non basta fare solo dichiarazioni, bisogna soprattutto promuovere interventi seri, a partire dell'Europa, che ad oggi ancora non ha posto in essere, ad esempio, quei princìpi di solidarietà in favore degli Stati che si trovano in situazioni di grave difficoltà, così come previsto dell'articolo 100 del suo Trattato istituivo.

vi è la necessità di incidere sotto il profilo del risanamento dei conti pubblici, con particolare riferimento al problema della riforma delle pensioni. Com'è noto, gli italiani lavorano da tre a poco meno di cinque anni in meno della media dei lavoratori europei. Ciò avviene perché si va in pensione da 1,3 a 2,3 anni prima rispetto alla media europea. Questo divario rispetto al resto dell'Europa provoca un incremento dei costi della previdenza italiana più alto del 4,4 per cento rispetto alla media europea e tocca il 14,7 per Non è peraltro accettabile che in Italia lavori solo il 19 per cento di coloro che hanno tra 60 e i 64 anni, mentre in Gran Bretagna sono il 50 per cento e in Spagna e Francia il 33

Non si può pensare che solo la politica dei tagli lineari serva al contenimento dei conti pubblici, ma vi è la necessità di riattivare circuiti virtuosi di razionalizzazione della spesa. Con riferimento al tema specifico del sostegno alla disoccupazione, i dati che, ad esempio, una recente ricerca del CERN evidenzia ci portano a ritenere che vi sia una stretta connessione con quella che abbiamo definito l'esigenza di un nuovo patto generazionale, che comporta la necessità, da un lato, di intervenire con politiche di sostegno al reddito delle famiglie, soprattutto quelle dei lavoratori precari,

9,2 miliardi nel 2010, 13,1 nel 2011, 16,3 nel 2012 e 18,8 nel 2013.

più concreto, l'introduzione di un sussidio unico garantito per tutti i disoccupati, indipendentemente dal tipo di contratto, che garantisca in partenza il 65 per cento della retribuzione precedente e non meno di 500 euro mensili,

seria ed equa riforma del sistema pensionistico, sia nella fase transitoria che nella fase di più lungo periodo. In questo contesto si può e si deve realizzare una politica che guardi ai lavoratori cosiddetti precari, posto che siamo in presenza di un fenomeno molto diffuso, che riguarda un lavoratore italiano su otto, di un fenomeno in crescita, e posto che si tratta di lavoratori privi di tutela molto spesso con famiglie da mantenere. Dobbiamo inoltre constatare, signora Presidente, che le misure che il Governo ha predisposto nel pacchetto anticrisi si sono in realtà rivelate non solo inefficaci nella sostanza, ma soprattutto ma soprattutto inadeguate a favorire le famiglie e le imprese che sono i soggetti deboli del nostro sistema, perché si sono rivelate misure *una tantum* e discrezionali e discrezionali non accompagnate da una visione strategica dei provvedimenti e delle provvidenze da impiegare per uscire dalla crisi. Faccio un esempio: del

Se i genitori sono conviventi e non sposati, avranno diritto ad un *bonus* doppio perché nel caso di convivenza non vige il cumulo dei redditi, per le persone sposate invece sì;

vincolo contrattuale ed alcuna sanzione nel caso in cui il sistema creditizio non rispetti il cosiddetto codice etico e quindi non orienti il finanziamento e la spinta, il sostegno economico, nei confronti delle piccole e medie imprese e delle famiglie.

nella mozione presentata dai colleghi del Partito Democratico, in un contesto più ampio che preveda misure che secondo noi il Governo deve adottare, anche se nel breve periodo possono non essere compatibili con

Le sintetizzerò per avviarmi velocemente alla conclusione. Riguardano, in particolar modo, il sostegno reale alla famiglia con figli, con l'introduzione del contributo di 100 euro al mese per il primo figlio e 50 per ogni altro figlio per famiglie con un tetto di reddito familiare di 50.000 euro; forti iniziative che spingano le banche a concedere credito per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; un patto generazionale che implichi una tempestiva riforma, nel senso da noi indicato, del sistema previdenziale e degli ammortizzatori sociali e che tenga conto e riconosca alle donne lavoratrici, ai fini dell'innalzamento dei limiti pensionistici, dell'attività prestata a sostegno di anziani,

riassuntiva della nostra posizione su tutte le questioni riguardanti le politiche economiche e fiscali del Governo rispetto alle quali anche il sostegno alla disoccupazione diventa un tassello importante, ma non l'unico, per uscire dalla crisi.

Signor Presidente, non è la prima volta che in quest'Aula discutiamo della crisi economica, una crisi internazionale che ha il suo epicentro negli Stati Uniti e la cui ampiezza e profondità investe in misura pesante anche il nostro Paese. I dati più recenti diffusi dalla Banca d'Italia, da Confindustria, dal Consiglio europeo e, da ultimo, dall'INPS dimostrano che il Paese è ormai in piena fase recessiva. Le conseguenze di questa crisi sul sistema produttivo e sull'occupazione sono drammatiche. La produzione industriale diminuisce del 12 per cento. Si moltiplica il ricorso alla cassa integrazione (quella ordinaria registra un aumento del 500 negli ultimi due mesi, come riportano dati recentissimi dell'INPS, si è registrato un aumento dei disoccupati di circa 370.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. siamo in presenza di una crisi economica e sociale senza riscontri nella storia dell'Italia repubblicana, che richiede interventi straordinari per sostenere il lavoro e le imprese. Finora, invece, il Governo, anche con l'approvazione delle ultime misure, si è limitato a proporre interventi *una tantum* assolutamente insufficienti misure totalmente inadeguate, come quelle previste a sostegno delle famiglie e per i lavoratori precari. In sostanza, siamo in presenza di scelte legislative da parte del Governo che sottovalutano la gravità della crisi economica ed industriale in corso, che non intervengono con misure adeguate per salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori.

Da ultimo, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ammette a denti stretti che la crisi c'è ma aggiunge, subito dopo, che essa non avrà effetti negativi sul piano sociale. che la gravità della crisi in atto richieda un intervento strutturale, sostenuto da un piano finanziario significativo, come peraltro stanno facendo Paesi come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna. C'è bisogno di una riforma organica degli ammortizzatori sociali per garantire a tutti i lavoratori una tutela sociale adeguata; c'è bisogno di un innalzamento delle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro dipendente autonomo e da pensione per sostenere i consumi. Solo così, senatore Castro, si può sostenere l'economia: altro che misure novecentesche! Soprattutto (questa è una proposta che abbiamo formalizzato nella nostra mozione), è necessario approntare misure che assicurino forme di tutela economica tramite un assegno mensile di disoccupazione per quei lavoratori che, in caso di

questo provvedimento, perché, così come sono state reperite per interventi iniqui ed inefficaci, come l'abolizione dell'ICI, si possono reperire anche in questa fase, con una precisa volontà politica, naturalmente, attraverso altrettanto precisi interventi, come peraltro noi indichiamo nella nostra mozione a cui, come diceva ieri il nostro segretario Franceschini, si deve aggiungere un contributo straordinario di solidarietà a carico dei redditi più alti.

in maniera caricaturale la nostra proposta. Il Presidente del Consiglio, come abbiamo visto nei giorni scorsi, ha sostenuto che l'attivazione di un assegno mensile per i disoccupati favorirebbe i licenziamenti e il ricorso è del tutto evidente che si tratta di una risposta strumentale, assolutamente inaccettabile, che dimostra l'assoluta insensibilità e persino l'insofferenza nei confronti di chi vive del proprio lavoro.

onorevoli colleghi, vorrei tentare di rispondere a tre domande: perché siamo qui, questa mattina, a parlare di questi argomenti, di che cosa stiamo parlando in realtà e di che cosa dovremmo parlare e dovremmo essere chiamati a votare in quest'Aula. Perché ne stiamo parlando

Franceschini, la mattina, facendosi la barba e guardandosi allo specchio, ha detto: «Ohibò, c'è una grande crisi e allora diamo uno stipendio a tutti».

è chiamata a spendere tre ore di tempo su tale argomento. Seconda domanda: di che cosa stiamo parlando? Se leggiamo attentamente la mozione Franceschini (spero solo che la maggioranza dei colleghi senatori del Partito Democratico, che ha sottoscritto nella sua totalità quella mozione, non l'abbia letta e non sappia di che cosa stiamo parlando), presto detti: l'andamento della crescita economica nel 2008 è stato del meno 1 mezz'ora fa l'ANSA ha diffuso i dati sull'andamento dell'ultimo trimestre: meno 2,9 se si invertisse la tendenza nella seconda metà di quest'anno, nel 2009 avremmo meno 2,6 per cento e forse zero nel 2010. Faccio presente ai colleghi senatori che ogni 1 per cento in meno di crescita economica comporta circa 300.000-350.000 disoccupati in più. Questo è il quadro serio che abbiamo di fronte

la proposta della mozione si riferisce a chi perde il posto di lavoro dal 1° settembre del 2008 in poi,

con le stesse moltiplicazioni (uso le tabelline), altri 17 miliardi di euro, per un totale di spesa, in base a

dei quali stiamo parlando in quest'Aula. Francamente, stiamo perdendo tempo in demagogia irresponsabile. Se togliessimo da questi numeri i circa 500.000 disoccupati che non hanno mai lavorato, coloro cioè che sono in cerca di prima occupazione

a perdere tempo su queste tematiche, non per la gravità della situazione, ma per la demagogia delle proposte! *(Commenti è evidente - lo sanno tutti, in particolare gran parte dei miei amici e colleghi senatori del PD - che un provvedimento del genere sarebbe un'induzione a licenziare e ad accettare il licenziamento, perché è storia d'Italia; infatti, garantire un reddito in questo modo significa palesemente incentivare una connivenza tra imprese e lavoratori

vera logica perversa. La situazione della crescita e delle prospettive occupazionali è seria, ma qui dobbiamo scegliere la logica: provvediamo ad intervenire *ex post*, cercando di sostenere, come sacrosantamente si deve fare, coloro che perderanno il posto di lavoro con gli ammortizzatori sociali che il Governo sta approntando, oppure è più responsabile cercare di dirottare le risorse per sostenere le famiglie e le imprese per minimizzare quell'effetto negativo, per evitare

27 miliardi di euro sono più efficaci se assegnati a sostegno della famiglia, con uno schema di coefficiente familiare che parta dalle deduzioni per carichi familiari, figli e nonni; sono molto più efficaci per dimezzare l'IRAP a tutte le piccole e medie imprese; costerebbe lo stesso ammontare.

di maggioranza, Governo e opposizione è discutere su dove prendere tali risorse. Allora, francamente, come si dice al mio Paese, «mi calano le braghe», perché la copertura

questa è la copertura dei 27 miliardi della mozione proposta dal Partito Democratico. Francamente, io andrei invece a proporre delle coperture per uno stesso ammontare che riguardino gli sprechi dei 45 miliardi di fondi perduti in conto corrente e in conto capitale, gli sprechi del dilagare della spesa nel settore della sanità, nel settore degli acquisti della pubblica amministrazione, 40 miliardi in più in quattro anni. Lì il confronto politico dovrà diventare serio, prendere le risorse per poi, a mio parere, concentrarle a sostegno delle famiglie e delle imprese per evitare che la gran parte di quel milione di disoccupati in più che voi prevedete

non solo svolge un'azione economica di sostegno al ciclo, ma anche una grande azione di perequazione sociale mettendo al centro